al presidente Andreotti, che ieri ha compiuto gli anni, rivolgo un caloroso saluto da parte di tutti noi. Auguri, Presidente. La Conferenza dei Capigruppo ha ribadito la validità del calendario fissato prima delle ferie,

Per quanto riguarda la settimana successiva, allo stato c'è il ritiro della mozione di sfiducia presentata dai Gruppi dell'opposizione

Vescovo di Roma, ha rinunciato a pronunciare la sua *lectio magistralis* all'Università «La Sapienza» perché impedito da un'opinione creata ad arte da 67 persone che si chiamano professori. lui, professore universitario nonché Capo della Chiesa Cattolica, viene impedito di parlare all'Università di Roma «La Sapienza», fondata da un Papa.

dall'estrema sinistra all'estrema destra e in ognuna delle persone che la compongono, in nome del principio liberale della libertà di parola e di pronunciare un intervento magistrale in qualsiasi università in qualsiasi università del mondo per qualsiasi persona del mondo, segnatamente nell'università italiana che si chiama «La Sapienza» e non può chiamarsi intolleranza. Vorrei che ognuno di noi qui desse la sua testimonianza a fianco del professor Ratzinger, testimoniandogli la lealtà di questo Senato laico, da professori a professori, per la libertà di parola in Italia.

per la verità sgradita, alla ripresa dei lavori nell'anno 2008 che consiste nel non avere più a disposizione la rassegna stampa

dell'insegnamento e del ruolo della cultura. Piuttosto, è un'escrescenza, quella dell'Università di Roma, di un rigurgito giacobino e sessantottino. È inconcepibile che in questo Paese un intellettuale come Papa Ratzinger non possa prendere la parola all'Università di Roma. Penso che se al posto del Pontefice si fosse recato all'Università un

invece assistito ad un'esibizione muscolare di alcuni - dicono - insigni studiosi

nulla di più falso, perché il Pontefice in una sua nota, in verità, portava come esempio

Questo è un secolo di persecuzioni anticristiane: circa 300.000 cristiani tutti gli anni nel mondo vengono uccisi per motivi di odio religioso. È evidente che questo atto di violenza culturale fa il pari con quel clima di profonda intolleranza, ma nasce da un sottofondo culturale giacobino e neototalitario, in cui lo spazio per la tolleranza si è nettamente ridotto: è la vittoria del «politicamente corretto», la vittoria dell'individualismo, la vittoria di una certa ostentazione di un orientamento sessuale ben preciso. Presidente, siamo profondamente preoccupati siamo profondamente preoccupati e vorremmo che quelle frange politiche che, in qualche modo, fanno riferimento a settori di questo Parlamento, trovassero una profonda deprecazione ed una profonda condanna anche da parte di certi Gruppi.

Paese. Ritengo che qualche piccola spiegazione autocritica, anche fortemente autocritica, e richiesta di perdono il Pontefice le debba fare. Starà poi a tutti decidere se perdonarlo o no. *(Applausi dai Gruppi Presidente, su questa vicenda molto sgradevole riguardante la visita del Santo Padre all'Università di Roma, il mio contributo è quello di un professore di quella stessa università. Desidero informare i colleghi del Senato

Mi sembra incredibile che alcuni colleghi si siano arrogati il diritto di concorrere a impedire la parola. Questo gesto non fa onore a chi l'ha chiesto. Fa invece onore al Papa aver rinunciato alla parola in questo momento. Ribadisco che la questione, di estrema preoccupazione, mi induce a ritenere

In conseguenza di quanto è stato detto sulla decisione presa dal Pontefice Benedetto XVI di non partecipare all'inaugurazione dell'università di Roma, ritiro la mia proposta, che era quella di pregare il presidente Napolitano di inaugurare a sua volta i corsi dell'università Gregoriana. In ragione del fatto che Chiesa Cattolica e Stato italiano sono pari ciascuno nel suo ordine, mi sarebbe sembrato che questo scambio potesse ridurre

alcuni colleghi di quest'Aula - altri lo sanno perché ne abbiamo parlato in Commissione affari esteri - che questa mattina l'Ambasciatore di Israele si è recato nella sala stampa della Camera e con alcuni parlamentari, alcuni giornalisti italiani e alcuni parenti degli ostaggi, ha ricordato un problema che ormai sta diventando lungo anni: mi riferisco alla scomparsa nel nulla degli ostaggi israeliani, di cui non si hanno più notizie, né sul versante Hezbollah, né sul versante Hamas. Si tratta di tre giovani la cui vita è stata radicalmente oscurata dalla mancanza totale di contatti,

sia perché a noi stessi è stato chiesto aiuto dalle madri, dai padri, dai fratelli, dalle sorelle di questi ventenni scomparsi nel nulla,

(che a quanto risulta sono state frequenti, dato il ruolo che ha l'Italia in questo momento nell'area) per rompere questo silenzio, questo isolamento, questa gravissima e crudelissima condizione nella quale sono messi gli ostaggi e le loro famiglie.

dei parlamentari e della casta e che avevano indicazioni dal Ministero dell'interno di usare misure dure nei confronti dei manifestanti e ancor più

sono ogni mattina a disposizione dei cittadini e vigilano, svolgono il loro ruolo, che non è soltanto quello di legislatore. Si deve avere almeno il rispetto delle istituzioni.

Signor Presidente, non solo sono mortificato come senatore della Repubblica, oltre che come cattolico, per quanto è successo - ringrazio sua Santità che, con il suo atto di rinuncia all'invito a presiedere l'apertura dell'anno accademico alla Sapienza di Roma, ha voluto rasserenare gli animi

la pace fra lo Stato italiano e il Vaticano è stata foriera di momenti di grande attenzione reciproca ed ha soprattutto prodotto fatti positivi sotto ogni aspetto per quanto riguarda l'interesse dello Stato.

non può finire con un solo annuncio in questa sede, ma deve avere un seguito fatto di chiarimenti per il bene del nostro Paese. La pace fra lo Stato italiano e la Chiesa di Roma è

come professore ordinario de «La Sapienza» giudico molto grave che il Santo Padre sia stato posto nelle condizioni di non poter intervenire all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università statale di Roma. Poiché Poiché esistono ragioni per ritenere che il Ministero dell'interno dello Stato italiano si sia dichiarato non in grado di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza in tale circostanza, giudico che la conclusione di questa triste vicenda rappresenti una sconfitta di quello Stato di cui facinorosi presumono di rivendicare l'autonomia e la sovranità rispetto all'autorità religiosa. *(Applausi dai

credo che una nazione in ostaggio di 67 individui beceri e intolleranti, cattivi maestri cresciuti nel brodo di cottura di un comunismo che ha intossicato la società italiana, debba fortemente reagire. Nel Paese delle moschee, della tolleranza verso tutto e tutti, ormai si è intolleranti solo nei confronti della Chiesa e della religione cattolica. Il Senato deve reagire con forza, signor Presidente. Noi senatori della destra chiediamo un suo passo ufficiale come seconda carica dello Stato. Stato. Il Senato deve reagire e stigmatizzare perché questo comportamento non solo ha mortificato una importante università come La Sapienza, ma ha anche offeso tutto il popolo italiano.

conoscendo la sua profondità di analisi e correttezza, perché si faccia interprete di un diffuso sentimento del Senato della Repubblica e stigmatizzi fortemente quanto è accaduto facendosi promotore affinché vicende analoghe non debbano più accadere. Era la gaffe

Il primo perché è una rinuncia a visitare l'università. Signor Presidente, colleghi, la cultura, l'università e la scuola sono i luoghi inclusivi, tolleranti ed aperti per definizione. Quando non hanno queste qualità non sono. Il secondo motivo che mi ha addolorato è che ciò sia accaduto con riferimento all'università di Roma. Roma è la città dell'accoglienza, capace nell'anno 2000 di essere la capitale dell'accoglienza del mondo. Roma ha ricevuto dalla Santa Sede e dal Papa i ringraziamenti più straordinari e credo più graditi per il grande lavoro di accoglienza che la città ha svolto nell'anno 2000, quando quasi 30 milioni di pellegrini sono venuti a visitarla. Che sia stata resa difficile, fino ad impedirla, la visita del Papa all'università, che sia stato usato come argomento Galileo Galilei, dimenticando che la Chiesa, contrariamente a quanto facciamo noi,

Papa. Pertanto, si esprime un profondo dispiacere per le ingiustificate critiche e censure all'invito del Santo Padre. Lalibertà di espressione deve prevalere su ogni forma di censura, che non ha niente a che fare con la libertà della ricerca. Anche noi ringraziamo la Santa Sede, come è già stato detto, per la forma in cui ha reagito. Vuole soprassedere sull'invito stesso e con questo atto ha anche palesemente

direzione. Al senatore Colombo comunico che accetto il suo invito, comprendendo il dramma e la grande questione della scomparsa dei tre giovani. Quindi, mi rapporterò con il Governo per sottolineare la necessità di un impegno continuo.

Conosco anch'io l'università «La Sapienza», non come insegnante ma come allievo - ahimè - di tanti e tanti anni fa,

tra le aziende sanitarie e le università, venga in discussione proprio il giorno in cui abbiamo ricordato la funzione e la grandezza dell'università come luogo di incontro e di confronto. Quindi, prima di leggere la relazione, voglio associarmi al dispiacere profondo per la condizione di intolleranza, di cui si è fatta oggetto la università «La Sapienza». Me ne dispiace molto. Il disegno di legge in esame reca vari interventi nei settori sanitario ed universitario, intesi ad assicurare sia la completa integrazione fra l'attività didattica e di ricerca delle facoltà di medicina e chirurgia e l'attività assistenziale, sia la piena funzionalità del Servizio sanitario nazionale. L'integrazione è necessaria sia per la formazione dei professionisti di nuova generazione che per una migliore sanità sul piano nazionale. La costituzione dell'azienda integrata, ospedaliero-universitaria risponde a criteri di ottimizzazione delle tre funzioni: didattica, ricerca, assistenza, nel pieno rispetto dei relativi profili professionali e nella prospettiva di un miglioramento delle diverse funzioni fino al raggiungimento dell'eccellenza. L'articolo 1 prevede la costituzione dell'aziende integrate ospedaliero universitarie. Le disposizioni sono, in particolare, volte a concretare il "modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria", stabilito dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, modello che, in genere, non è stato ancora attuato. Dall'intervento normativo sono, di conseguenza, escluse le aziende già costituite, in base a disposizioni regionali, secondo il suddetto modello. Nelle aziende integrate confluiscono le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, le aziende ospedaliere integrate con l'università, i policlinici universitari di diritto pubblico a gestione diretta, i presìdi ed aziende ospedaliere nei quali insista la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché gli altri soggetti di diritto pubblico operanti in ambito ospedaliero-universitario. Si segnala inoltre che il comma 3, inserito dalle Commissioni riunite 7a e 12a, disciplina i protocolli d'intesa con le università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari. Nell'articolo 2, comma 1, che concerne gli immobili in uso alle università statali per le finalità istituzionali delle facoltà di medicina e chirurgia, si dispone il trasferimento a titolo gratuito alle università della proprietà dei suddetti beni, qualora essi appartengano al patrimonio indisponibile dello Stato, e la concessione in uso gratuito alle medesime, qualora i beni facciano parte del demanio statale o sia in corso una verifica sull'interesse culturale degli stessi. La concessione in uso gratuito è attribuita fino alla permanenza dell'impiego istituzionale del bene; il concessionario esercita il diritto di proprietario e ne assume gli oneri, nei limiti imposti dalla natura demaniale del bene. Nell'ipotesi summenzionata di verifica in corso dell'interesse culturale, l'esito negativo della stessa determina il trasferimento della proprietà del bene all'università. Lo stesso comma 1 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le università e l'Agenzia del demanio redigano i verbali di consistenza, i quali costituiscono titolo per la trascrizione (della proprietà o della concessione) da parte delle stesse università, eseguibile "senza oneri, diritti o tributi". Il comma 3 estende le disposizioni dì cui al precedente comma 1 ai beni immobili la cui proprietà sia stata già trasferita dallo Stato alle università statali, per le loro finalità istituzionali. Il comma 4 prevede che, entro trenta giorni dalla trascrizione summenzionata, le università statali concedano in uso gratuito alle aziende integrate ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 1 i beni immobili di cui siano proprietarie, ovvero concessionarie, e che questi siano già adibiti ad attività assistenziali collegate alle attività istituzionali delle facoltà. Secondo le previsioni aggiunte dalle Commissioni riunite 7a e 12a, gli immobili in esame oggetto di trasferimento alle università sono inalienabili; i beni demaniali di cui al presente articolo non possono essere impiegati per fini lucrativi e i beni, mobili ed immobili, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale hanno il vincolo di destinazione alla medesima. L'articolo 3 disciplina le procedure di verifica dell'attuazione dei precedenti articoli 1 e 2, procedure che, nel testo approvato dalle Commissioni riunite, sono affidate alle Regioni e alle Province autonome, anziché ai Ministeri competenti. Stante però il parere negativo della 1a Commissione, dal momento che l'emendamento attribuirebbe poteri sostitutivi alle Regioni in un ambito che coinvolge attività e competenze delle università, e conseguentemente competenze dello Stato, si propone di tornare alla versione originaria del disegno di legge e di affidare la verifica dello stato di attuazione delle norme prioritariamente ai due Ministeri di competenza, che ovviamente dovranno sentire le rispettive Regioni. L'articolo 4 dispone uno stanziamento uno stanziamento ai fini dell'istituzione, in ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda integrata ospedaliero-universitaria ed istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'unità di gestione del rischio clinico.

Nell'ambito del mercato del lavoro, il comma 1 elimina il divieto alle università pubbliche e private di svolgere attività di intermediazione in forma consortile, a condizione che queste vengano svolte senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo dell'interconnessione alla Borsa continua nazionale del lavoro, nonché dell'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del suddetto mercato. Il comma 2 allinea la durata dell'incarico dei direttori dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza a quanto previsto dal decreto che regola i criteri dell'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistico-musicali in materia di elezione dell'organo direttore di tutte le istituzioni di alta formazione artistico-musicale. Viene data così applicazione anche per le due Accademie sopramenzionate al sistema ordinario di elezione dell'organo in questione, facendo cessare il tempo indeterminato per la durata dell'incarico.

L'articolo 7 (introdotto dalle Commissioni riunite 7a e 12a) consente una forma di ammissione in soprannumero alla formazione specialistica per i soggetti già in possesso del titolo di specialista. La metà dei posti in soprannumero è riservata al personale medico di ruolo in servizio negli ospedali pubblici, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in strutture assistenziali identificate nei protocolli d'intesa fra università e Regione o in altre strutture assistenziali a tal fine indicate dalla Regione. infine, si riferisce alla convocazione delle organizzazioni sindacali. Poiché le aziende integrate ospedaliero-universitarie vengono a configurare una realtà nuova e già di per una realtà nuova e già di per sé molto complessa, si ritiene più opportuno non inserire cambiamenti nelle convocazioni sindacali, per cui ho presentato un emendamento volto alla soppressione dello stesso articolo.

è abbastanza ovvio), in quanto con esso stiamo cercando di integrare il più possibile l'attività didattica e di ricerca dell'università con l'azione assistenziale del Sistema sanitario nazionale.

sono presenti in disegni di legge già annunciati direttamente dal Ministro. Quindi, a mio avviso, stiamo creando delle sovrapposizioni. Le famose aziende integrate le vogliamo tutti. L'unica differenza che avverto, per il momento, nel testo (e non so cosa accadrà con gli emendamenti) è che, nonostante i vostri grandi annunci di pari dignità per tutti, per l'alto ruolo che svolgono le università e le strutture non solo pubbliche o prettamente pubbliche, ma anche quelle, diciamo così, private, ma in realtà condotte dalla Chiesa, che

dopo averlo annunciato, dopo aver addirittura parlato di ingenti finanziamenti, siate coerenti. Ci riserviamo pertanto di dare un giudizio al termine dell'esame

di proprietà del demanio possa essere dato una volta per sempre (con tutti i limiti, con tutti i paletti necessari per questa funzione) alle università e agli ospedali per esplicare questa funzione. È una cosa, a mio avviso, ovvia e necessaria, ma era urgente a luglio ed oggi è già stata superata da altri provvedimenti. Quindi, fortunatamente, alcune strutture stanno già operando e, essendo entrate direttamente in possesso di queste strutture, stanno operando anche delle ristrutturazioni.

solo parzialmente su problemi parziali; essa non risolve niente e fra qualche giorno verrà superata da ciò che avete già enunciato. È anche da voi enunciato ha dei ritardi spaventosi se è vero che parlavamo di questa legge a luglio e la stiamo realizzando a gennaio! Vi chiedo: è possibile che il Governo italiano debba proseguire con questa miriade di leggi che creano soltanto confusione? Se sullo stesso provvedimento

stiamo parlando di una legge che dovrebbe concretizzare un decreto-legge del 1999 che non è stato mai realizzato e che con essa non riceverà nemmeno una carezza né una spintarella per muoversi. Ecco perché vi chiedo, per cortesia, per essere all'altezza del nostro ruolo, di parlare di cose serie: ci confrontiamo, ci scontreremo, ma parliamo di cose serie, non di leggi farsa o di enunciazioni che non servono a niente. *(Applausi dal

ha consentito di dare ancora maggior puntualità ad un intervento urgente e necessario per assicurare un efficace governo del nostro sistema di formazione dei medici. Il rapporto tra formazione dei medici e attività clinica e lo sviluppo e il ruolo che i policlinici e le strutture ospedaliere collegate alle università svolgono nel nostro sistema sanitario nazionale necessitavano di una revisione, che si ponesse a conclusione del percorso avviato nel 1999 con il decreto che istituiva le aziende ospedaliero-universitarie. Didattica, ricerca e assistenza sono tre funzioni già di per sé molto complesse, che abbisognano di un modello unico nazionale per la loro necessaria integrazione. Senza ledere l'autonomia di cui sono dotate le università e senza porre in discussione il ruolo delle Regioni, si è voluto quindi dare un'indicazione normativa precisa per un modello organizzativo che già ha dimostrato, sperimentalmente in alcune Regioni, la propria efficacia. In ragione di questa decisione, è quindi possibile definire con maggior puntualità i diritti sul patrimonio immobiliare da parte delle aziende ospedaliero-universitarie. Esso dovrà essere inalienabile e mantenere una chiara destinazione d'uso. Questa soluzione consentirà di accelerare quegli interventi utili a rendere più efficienti le funzioni didattiche e ospedaliere che si svolgono in quelle sedi. Il provvedimento in discussione fornisce finalmente risposte adeguate alle domande organizzative del nostro sistema sanitario e consente di affrontare in modo più equilibrato

È evidente come il nostro sistema sanitario, che pure è una delle punte avanzate del *Welfare*, non goda dell'attenzione dell'opinione pubblica per i tantissimi, quotidiani esempi di eccellenza, ma ben più spesso per eventi drammatici, legati ad errori umani. Esistono ormai consolidate procedure e modelli organizzativi capaci di ridurre significativamente quegli errori: indicare questa come una priorità che richiede investimenti è un segnale positivo per il rispetto della salute dei cittadini, che devono potersi affidare con serenità al nostro sistema sanitario nazionale. Certamente, nel provvedimento esistono alcuni aspetti che avrebbero meritato una riflessione più approfondita e che ci auguriamo nei prossimi mesi possano essere oggetto di interventi efficaci: da un lato, il processo di precarizzazione (al quale anche in quelle aziende ospedaliero-universitarie assistiamo) e, dall'altro, la qualità della formazione e il rigore nella selezione dei futuri medici. A fianco alla piena applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo del 1999, sarebbe utile ragionare di come la specificità formativa degli ospedali di insegnamento possa essere ulteriormente valorizzata, con la consapevolezza che queste strutture sono fondamentali per lo sviluppo di una futura classe medica capace ed efficiente. Pensiamo, ad esempio, alla gestione degli specializzandi, che, troppo spesso risultano essere manovalanza a basso costo e non professionisti in formazione. Il passaggio da borse di studio che non garantivano alcun diritto alle nuove configurazioni previste dall'ordinamento ha consentito di migliorare lo stato delle cose, ma le recenti proteste di questi medici in formazione ci sollecitano ad affrontare rapidamente questo elemento di disagio. E ancora non si è affrontata la grande questione dell'accesso alle scuole di specializzazione. Così come resta aperto il tema del reclutamento di docenti e ricercatori e quello della qualità delle attività didattiche nel corso della specializzazione. Spero che dopo questo primo provvedimento sapremo celermente affrontare il tema dell'accesso alle scuole di specializzazione: la definizione in sede locale delle graduatorie, troppo spesso ha significato graduatorie incomprensibili, in spregio ad un rigoroso principio meritocratico. Negli altri Paesi la scelta di un concorso nazionale, dove i primi in graduatoria hanno la possibilità di scegliere le migliori scuole di specializzazione, garantisce maggior trasparenza e assicura lo sviluppo di grandi scuole mediche. Per ora ci avviamo a regolare un aspetto, pur importante, che riguarda chi, già medico specialista, voglia ottenere la seconda specializzazione. Un scelta utile che consente di migliorare le competenze di chi già opera, ad esempio, in ambito ospedaliero, senza togliere opportunità ai giovani laureati. Così come sarebbe utile fare chiarezza sul passato, restituendo certezza a chi abbia svolto l'anno scorso l'esame di specializzazione e che per un elemento tecnico, come la discrasia tra ingresso in specializzazione e abilitazione, oggi dovrebbe ripetere un esame già svolto con profitto. Ma permane la necessità di un intervento più complessivo, che faccia tesoro dell'esperienza maturata con i ricercatori nell'università. Per quanto attiene all'articolo 5, credo sia necessario un approfondimento sulla scelta dì favorire l'attività consortile di intermediazione per l'accesso al lavoro da parte di una varietà di enti pubblici e privati: non solo università, ma anche enti locali, scuole, associazioni imprenditoriali e camere di commercio. Dopo alcuni anni dall'applicazione della legge n. 30 del 2003, da cui origina questo strumento, credo che una riflessione sulla necessità

che il Governo ha già ripetutamente dichiarato di voler modificare, cioè il sistema disposto dalla citata legge n. 30, ci chiediamo se sia utile introdurre in questa sede un intervento così puntuale in un contesto che sta cambiando molto repentinamente. Non si tratta solo di un piccolo dettaglio, ma della funzione che si immagina per l'università, cioè se essa debba essere prioritariamente orientata all'attività di promozione professionale o all'attività di ricerca, e dove sia il punto di equilibrio tra queste due funzioni parimenti importanti. Così come, forse, la costruzione delle banche dati può essere un servizio utile agli studenti, altre attività della gestione di intermediazione sono assolutamente incoerenti con la missione dei luoghi della formazione: è evidente come si sia voluto stiracchiare un istituto concepito per altre istituzioni, e rafforzare l'errore non è forse la scelta migliore. Per questo abbiamo ripresentato, insieme ad altri colleghi, in Aula un emendamento che ci auguriamo possa trovare il consenso del Governo Per concludere, quindi, salutiamo con soddisfazione, nonostante alcune perplessità che spero riusciremo a correggere, questi interventi, ulteriormente migliorati dal lavoro delle Commissioni, ma speriamo che, sul nesso delicato tra sistema sanitario e sistema della formazione universitaria, questo sia un primo passo che rapidamente sapremo integrare con nuove e puntuali iniziative.

La mancata adozione del decreto che doveva mettere a regime il sistema di costruzione delle aziende

con un provvedimento per buona parte condivisibile ma che ci induce a sostenere alcuni emendamenti.

che, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, non assumono più natura vincolante per le Regioni in quanto la relativa disciplina deve essere ricondotta alla competenza regionale.

imprescindibile, anche se in proposito la Lega ha in mente una riforma che proporrà nella prossima legislatura (l'avevamo nel cassetto, ma purtroppo non vi erano risorse per attuarla nella scorsa legislatura)

indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 che, a seguito della riforma del Titolo V, sono stati riconosciuti dalla stessa Corte costituzionale non vincolanti per le Regioni. All'articolo 2 proponiamo di introdurre un vincolo di destinazione per gli immobili del patrimonio indisponibile dello Stato trasferiti in proprietà alle università perché crediamo che nel momento in cui lo Stato conferisce degli immobili debba anche non vorremmo trovarci un giorno con la sorpresa di destinazioni non propriamente congrue. All'articolo 4 riteniamo di ripensare la disposizione volta a istituire in tutte le strutture ospedaliere apposite unità di gestione del rischio clinico

Regioni debbano adottare apposite linee guida di gestione del rischio a carattere organizzativo e funzionale terapeutico. Non vediamo come, in un momento di devoluzione

onorevoli colleghi, la ridefinizione del rapporto tra le università ed il Servizio sanitario nazionale è un problema davvero annoso. Altri colleghi e colleghe hanno qui

La discussione di questo disegno di legge è avvenuta su iniziativa del Governo: apprezziamo moltissimo che tale iniziativa, sia pur nata da una situazione di urgenza (quella posta, in particolare, dal Policlinico di Roma

dal disegno di legge, così come lo consegniamo all'Aula, è fondamentale rispetto ad una situazione di inazione che si era protratta per troppo tempo. Pensiamo anche che sia stato importante prendere le decisioni che sono state adottate e che suggeriamo al Parlamento in relazione sia al patrimonio, che ai poteri che vengono conferiti per la sua gestione e, soprattutto, per la sua manutenzione. I problemi gravi di urgenza e di emergenza che si sono posti sono infatti stati dovuti proprio alle difficoltà nell'assunzione delle decisioni e, in qualche caso, anche alle difficoltà connesse alla mancanza di fondi. Ho espresso un giudizio positivo sul provvedimento così come uscito dalla Commissione, pur ritenendo che esso sia ancora migliorabile. Penso, in particolare, ad una questione, che vorrei richiamare. Questo disegno di legge contiene all'articolo 5,

possano svolgere attività di intermediazione e di manodopera. Quello che la norma proposta prevede - mi riferisco alla disposizione contenuta nel testo pervenuto dal Governo - è che venga abrogato l'impedimento, introdotto nel 2004 dal precedente Governo, a svolgere tale attività in consorzio. pari di altre forze della sinistra, abbiamo presentato emendamenti già in Commissione, ritenendo non comprensibile, ma anche politicamente sbagliato, attenuare i pochissimi vincoli esistenti sull'attuale sistema di deregolamentazione e di privatizzazione del collocamento. Dei due emendamenti che discuteremo successivamente, il primo è seccamente abrogativo, lasciando le cose come stavano, mentre il secondo limiterebbe l'azione di questi soggetti unicamente all'orientamento finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro (esso è anche quello che meglio esprime la posizione di cui siamo portatori). Devo aggiungere che in Commissione altri colleghi della maggioranza, così come lo stesso Governo, hanno avuto un atteggiamento in qualche modo incoraggiante. Riteniamo quindi che la ripresentazione in Aula di questi due emendamenti possa portare il Governo a riconsiderare una posizione, per altro anche contraddittoriamente espressa in due occasioni nella discussione in Commissione, in modo da evitare una distinzione all'interno dell'Unione su un punto delicato. Ricordo inoltre che tale punto è stato trattato dal programma dell'Unione

che fanno pratica e lavorano all'interno di quelle strutture. Eppure questi medici per anni sono stati dimenticati dal Servizio sanitario nazionale e dalle università. Se costoro avessero abbandonato tutti insieme e contemporaneamente il servizio che svolgevano, ci saremmo trovati improvvisamente senza il sistema d'emergenza dei policlinici universitari sull'intero territorio nazionale. Ma questo disegno di legge presenta anche un altro problema.

ad essere uno dei punti rilevanti delle contrapposizioni all'interno dei policlinici universitari. Quando si deve procedere alla nomina dei direttori generali dei policlinici, non è possibile prelevare un direttore generale da un'azienda dell'emergenza sanitaria (per il Lazio, faccio l'esempio del Policlinico Sant'Andrea, dove opera la seconda facoltà di medicina dell'università «La Sapienza») e catapultarlo in

l'intera università «La Sapienza» è in contrasto netto con il direttore generale nominato dalla Regione Lazio, il dottor Montaguti, il quale è diventato nemico delle organizzazioni sindacali al punto che il professor Frati è riuscito a farsi rieleggere un'altra volta preside della facoltà di medicina, aumentando addirittura i voti

quasi totalità dei docenti della prima facoltà di medicina proprio perché Montaguti in questi anni ha distrutto il sapere all'interno

insieme alla consorte dall'università. Quando ho fatto la somma dei due stipendi, mi sono accorto che Montaguti percepisce più di ogni altro professore universitario e docente. Montaguti ha partecipato anche alla gara per essere titolare di cattedra all'interno del Policlinico mentre ne è il direttore generale. Il Servizio

dei Ministri della salute e dell'università sarebbe quindi da gettare completamente alle ortiche, perché ancora una volta non risolve a fondo il problema.

La nostra università e le nostre facoltà di medicina ci sono invidiate dagli altri, ma non certo dalle Regioni e da chi sceglie i direttori generali.

onorevoli colleghi, la medicina universitaria è certamente nel nostro Paese una medicina di grande qualità. Tuttavia, ritengo che con questo provvedimento si rischi di appiattire la medicina universitaria sul Servizio sanitario nazionale. Si riduce, a mio avviso, il valore della componente di ricerca e didattica. Questo appiattimento si realizza proprio quando in tutto il mondo la ricerca biomedica è di punta, è al centro dell'attenzione di ogni Governo. Credo che un provvedimento, come quello che abbiamo che abbiamo oggi all'attenzione, intacchi gravemente l'autonomia universitaria perché le strutture ospedaliere universitarie sono messe sotto il controllo degli assessori regionali.

Abbiamo d'altro canto assistito, proprio nelle scorse settimane, allo scandalo della Liguria, dove i dirigenti delle strutture complesse erano stati lottizzati secondo logiche politiche dalla maggioranza al Governo in quella Regione. Lo stesso presidente della Regione, Burlando, ha dovuto giustificarsi pubblicamente per alcuni gravi episodi di malcostume che sarebbero stati denunciati proprio dai *media*. Ebbene, credo che la politica debba stare fuori dall'università e sarebbe dunque un errore approvare un provvedimento di questo tipo che confonde e riduce l'autonomia del nostro sistema universitario proprio in un settore strategico come quello della medicina. Devo anche aggiungere che ho parlato con molti docenti, con qualche rettore ed ho notato una forte contrarietà a questa misura. Mi chiedo allora se vi confrontiate con il mondo della ricerca. Il Governo non ha purtroppo l'abitudine di confrontarsi con il mondo della ricerca. Ancora una volta, caro ministro Mussi, lei esce perdente da un confronto politico: l'università esce umiliata e penalizzata. Potrei fare tanti nomi di docenti che mi hanno scritto e contattato in questi giorni, ma evidentemente a lei Ministro ed a lei, Presidente Prodi, non importa molto di tutto questo.

È un emendamento che riprende tra l'altro una battaglia che noi di Alleanza Nazionale abbiamo condotto nei mesi scorsi per consentire ai giovani laureati in corso di poter affrontare ed iscriversi alla specializzazione, ancorché non avessero sostenuto l'esame di abilitazione. Per quest'anno, nonostante l'originaria contrarietà del ministro Mussi,

fa ben comprendere come non vi sia molta materia, molta carne al fuoco, per quanto riguarda il sistema universitario. Eppure, come ha poc'anzi detto il collega Valditara, il Governo non rifugge mai dalla tentazione di mettere le mani dentro il sistema, non dimostrandoci mai qual è la logica che sorregge i ragionamenti o le iniziative. Non riusciamo mai a comprendere quale sia il disegno complessivo del Governo per l'università, perché esso interviene sempre in maniera episodica, per piccoli tratti, come ha fatto anche asservendo al sistema sanitario nazionale anche il campo medico accademico ed applicando a questo settore delicato e importante del nostro sistema universitario le regole tipiche della politica; quindi, dobbiamo pensare, anche della lottizzazione politica. Affidiamo alle Regioni ed al ragionamento delle politiche regionali quelle che dovrebbero essere strategie complessive della nostra eccellenza universitaria. Interveniamo

mi sembrava di intuire che grande spazio, grande attenzione e quindi grandi e importanti decisioni avrebbero atteso il settore universitario e della ricerca del nostro Paese. Pensavo che la coalizione e il Governo esponenziale di tale coalizione avessero su questo tema speso molto in termini di risorse e di impegni. Quindi, ho affrontato l'impegno in 7a Commissione con grande passione. La passione è andata però via via scemando, man mano che

quasi impotenti rispetto a scelte di cosiddetta maggioranza. Ricordo ancora nelle prime sedute il Ministro

Invece, andando avanti, assistiamo non solo a un ritardo dei finanziamenti, ma all'assoluta mancanza di un piano strategico per l'università. Continuiamo ad assistere a interventi non solo frazionati ed episodici, ma per nulla riferiti ad un disegno complessivo. Le università quotidianamente ci ricordano che ci sono i concorsi che devono essere banditi. Il mondo accademico ce lo chiede. I nostri ricercatori sono i peggio pagati. I nostri giovani nelle nostre università non si sentono protagonisti del sistema, non si sentono partecipi di un loro percorso di formazione. Tutto ciò in un momento in cui quotidianamente i mass media non fanno altre che denunciare il nostro essere fanalino di coda rispetto a tutti i Paesi europei. Il nostro sistema universitario e della ricerca è messo sotto accusa e in ogni caso siamo considerati il fanalino di coda. Ancora oggi, leggendo il «Corriere della Sera», ci troviamo di fronte alle statistiche, purtroppo negative, in cui eccelliamo a livello

con i fallimenti clamorosi di questo Governo nelle politiche sociali, con la diffusa decadenza amministrativa e con la perdita di autorevolezza assoluta di questo Governo,

Il Governo in questo caso sta fallendo su un aspetto fondamentale che riguarda la vita di una Nazione, quello della prospettiva, del futuro.

ricerca, che non investe nella capacità competitiva del proprio sistema (e la ricerca e l'università sono fattori fondamentali per la crescita della competitività) crea naturalmente nelle aspettative del Paese e nelle valutazioni che del Paese fanno tutti gli organismi internazionali un grosso *gap* negativo. Vi è poi un altro binario

di non essere competitivi rispetto ai coetanei europei, rispetto alla formazione degli altri giovani che matura in maniera maggiore rispetto alla propria. quando un Governo riesce ad uccidere anche la speranza, si tratta di un Governo che davvero fa male. Perché uccidere la speranza dei giovani, delle nuove generazioni, è davvero delittuoso, il segno di chi non si pone il problema, di chi non si sente addosso la responsabilità della crescita del Paese, ma soltanto il piacere del mantenimento della propria posizione di potere, della propria poltrona.

passando le decisioni fondamentali del settore accademico ai settori della politica regionale, mi sembra che, ancora una volta, possa consentirci di denunziare un'assoluta mancanza di strategicità. Cosa dobbiamo aspettare ancora perché il ministro Mussi, perché questo Governo ci sottoponga un piano di rilancio della nostra politica universitaria? Cosa dobbiamo ancora aspettare perché questo Parlamento possa trasmettere ai giovani del nostro Paese una parola di speranza? Cosa dobbiamo aspettare per limitare la perdita delle nostre migliori intelligenze a vantaggio di altri Paesi del Pianeta? Cosa dobbiamo aspettare ancora, sottosegretario Modica, per ottenere la possibilità di discutere in termini concreti di strumenti della nostra competitività complessiva? Il provvedimento non merita certo una riflessione così ampia, ma siamo indotti a farla proprio per richiamare il Governo a queste problematiche. Al relatore Fontana e ai membri della 7a Commissione permanente dico che non possiamo assumerci la responsabilità, da parlamentari, di non essere noi,

Troppo spesso i compromessi con la vostra coscienza diventano connivenza! Voi siete titolari, come membri di questo Parlamento, dello sfacelo che questo Governo sta consumando nelle nostre università e nel settore della ricerca scientifica. Cari colleghi, sarete voi, coloro che voteranno gli emendamenti e il provvedimento complessivamente, ad accreditarvi come titolari

Questo settore necessita davvero di campi larghi e di tempi lunghi. È però anche vero che, quando il campo si allarga e i tempi devono essere necessariamente lunghi per raggiungere i risultati, bisogna avere chiarezza di idee e di impostazione. Voi mostrate confusione,

in qualche modo, riflettono la complessità del disegno di legge che stiamo trattando. È vero che il riferimento alla legge n. 517 del 1999

non può che concorrere ad un miglioramento dell'assistenza, ma anche a un miglioramento della qualità dei processi decisionali.

all'università significa semplificare quei processi decisionali che possono condurre ad attivare quelle iniziative di miglioramento e di adeguamento delle strutture, affinché queste, a loro volta, rispondano sempre meglio ai fini istituzionali che la legge si propone. Certamente, anche questo è un punto di difficile attuazione. Questo disegno di legge offre una semplificazione dei processi decisionali che si può convertire in un miglioramento.

ma è anche vero che porre al centro dell' attenzione la qualità della sanità e la sicurezza del paziente rappresenta per l'istituzione assistenziale il più alto degli obiettivi da raggiungere. Infine, un passaggio interessante è quello che si riferisce alla formazione del personale già presente nelle università e anche nelle aziende ospedaliere, esso possa accedere, attraverso la possibilità di iscriversi a scuole di specializzazione, ad un aggiornamento del profilo professionale di quanto essi già fanno a quanto richiesto dal modello culturale di ciò che, in qualche modo, dovrebbero sapere. Tutto ciò rappresenta, a mio avviso, una puntualizzazione precisa e rigorosa di alcuni aspetti. Non sarà la cura solo di questi punti a migliorare *in toto* il sistema della sanità, ma sicuramente l'azienda integrata del policlinico-università potrà avvantaggiarsene. Certamente, nulla sostituisce la buona volontà e la decisione di assumere in prima persona la responsabilità di dare alla nostra sanità una svolta alta e forte e, nello stesso tempo, di acquisire dall'interno la consapevolezza che la qualità dell'assistenza non può guardare ottimisticamente al futuro se non è supportata da una qualità della ricerca.

gesto di riflessione, rielaborazione e miglioramento della qualità dell'assistenza. Mi auguro davvero che questo disegno di legge, grazie anche ad alcuni emendamenti che discuteremo domani, possa raggiungere sempre meglio i propri obiettivi profondi e, in questo modo, rispondere a quell'unico obiettivo, veramente

apparentemente di piccolo impatto, ma che in realtà era atteso e che riteniamo molto importante. Intervengo solo su un aspetto, rimandando rimandando agli interventi dei relatori per le altre osservazioni, che condivido perfettamente. Di fronte alla preoccupazione espressa da alcuni senatori, vorrei rassicurare che questo provvedimento va nella direzione di potenziare la presenza universitaria della didattica e della ricerca nel sistema sanitario nazionale. Non togliamo niente a nessuno. Anzi, diamo possibilità in più, più, un quadro di governo delle aziende migliore e, per la prima volta, attuazione ad una previsione, ormai di otto anni fa, che riteniamo particolarmente importante. Si tratta di quella che vede come poli di eccellenza del sistema sanitario nazionale pubblico le aziende ospedaliero-universitarie integrate, laddove si integrano la didattica, la formazione e la ricerca a più alto livello con l'assistenza a beneficio dei cittadini.

dava spazio prioritario naturalmente agli universitari, che hanno questo tra i loro compiti, ma anche a quella grande capacità di formazione e di ricerca presente nel servizio sanitario nazionale, nelle aziende integrate. rende possibile finalmente superare quelle contrapposizioni di cui qui ho parlato, per arrivare ad un sistema sanitario che risponda alle esigenze dei cittadini. Sembrano interventi di piccola portata: si parla di edilizia, di manutenzione, di nomine dei responsabili delle strutture. Sembrano piccole questioni, ma sono quelle che riescono a far venir fuori dalla secca dove si era incagliata negli ultimi anni la riforma del 1999, per darle completa attuazione. Lo ribadisco: tutto ciò rientra nell'ottica di un servizio sanitario nazionale pubblico che si arricchisce del contributo di alta formazione e di ricerca che viene dalle università e dal personale del servizio sanitario nazionale che lavora nelle aziende integrate. Va detto con chiarezza, perché penso sia un punto di successo del nostro Governo.